Signora Presidente, colleghi, come già detto molte volte ieri, siamo al decimo decreto-legge per quanto riguarda questa realtà industriale importante per il nostro Paese. È importante anche l'attività lavorativa che sta dietro all'impresa ILVA; allo stesso tempo, come più volte si è detto, bisogna salvaguardare l'ambiente e la salute di chi ci lavora, oltre che l'impresa, che ha un grande indotto sul territorio. Bisogna salvaguardare il Meridione. L'ILVA ha una sua concentrazione massima a Taranto, ma è diffusa anche in altre località come in provincia di Alessandria e Genova. Per cui, è sicuramente importante salvare questa impresa. Il punto è che probabilmente con questo decimo decreto forse i tempi sono stati un po' troppo dilatori.

Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, ho poco tempo disposizione - giusto cinque minuti - e non è semplice per me, come per altri, argomentare sufficientemente bene le mie conclusioni su un provvedimento che investe l'ILVA e il suo diretto sinonimo, la città di Taranto. La fiducia in questo senso non ci aiuta e rende ancora più stringente la necessità di fare sintesi. sintesi. Superata la discussione sulla costituzionalità o no del ricorso all'ennesimo decreto-legge sullo stesso argomento, qui c'è un dato, anzi un fatto, che ci deve far riflettere prima e che suggerisce, in modo più che evidente, come la decretazione di urgenza con l'ILVA alla fine non funzioni. Richiamando altri momenti di discussione sui vari decreti proposti nel passato, intendo ribadire che anche questo provvedimento evidenzia in tutta la sua potenza la crisi dell'ILVA e il rincorrersi di continue soluzioni tampone, perché forse manca una visione strategica o - se si vuole pensare positivo - perché non si riesce ad esplicitarla e a portarla avanti.

nell'inquinamento del suo territorio. Questo decreto-legge - lo hanno ricordato in tanti - è l'undicesimo provvedimento che riguarda per materia l'ILVA, ma, come in una tragica sintesi tra gli sforzi di Sisifo e il lavoro di Penelope, ci troviamo sempre allo stesso punto, spostando magari un po' più in là le scadenze e le proroghe, concedendo o estendendo qualche guarentigia in più a commissari o possibili acquirenti. Condivido dunque lo sforzo di mantenere salda la convinzione che la vendita dello stabilimento, al di là del rappresentare la volontà di continuare a produrre acciaio in un territorio ferito, rappresenta la volontà di non chiudere immediatamente un'industria che dà occupazione. Dobbiamo quindi leggere il decreto-legge come uno strumento per dare stabilità agli investimenti dei privati che rileveranno lo stabilimento e che, nel contempo, creeranno quella situazione solida in cui le strategie di ambientalizzazione trovano concretezza e attuazione. Ecco allora giustificate e anche giustificabili le variazioni al piano da parte dei privati che acquisteranno, perché in tal modo si avvieranno le strategie vere per la ricostruzione di Taranto, fermo restando però che l'obiettivo finale sarà quello di offrire un diverso futuro alla città ionica, che discuteremo con la gente e la città, e di cui il patto per Taranto, firmato dal Presidente del Consiglio, rappresenta solo un'anticipazione di ciò che il Governo deve fare per essa. Perché l'ordalia messa tragicamente in essere tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro - l'ILVA e Taranto rappresentano questa drammatica sintesi - non può essere affrontata e tantomeno risolta solo a colpi di decreti-legge e ancor di più a colpi di cieca fiducia. Perciò, rientrando nelle maglie del decreto-legge in votazione, non posso non rilevare come questo provvedimento non si discosti poi molto dai precedenti anche se, per onestà, si possono cogliere dei timidi passi in avanti,

confermiamo invece che occorre dare spinta alla sua attuazione, per dare risposte alla sofferenza di una città aggredita sotto il profilo ambientale. ulteriore riserva era stata espressa circa l'eventualità di rendere possibile una modifica dell'AIA, anche se ora si registra una ulteriore novità: Riscontro infatti un parziale ascolto, come per Arpa, ad alcune criticità poste in passato, ad esempio laddove si individuava il DPCM come strumento di autorizzazione che "tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale".

Il provvedimento è sbagliato e non tutela l'ambiente. Signori colleghi, il nostro Gruppo, già in occasione del nono decreto ILVA, aveva fatto notare in quest'Aula come la linea indicata dal decreto-legge non fosse affatto la soluzione magica, capace di dissipare tutte le ombre legate alla faccenda come sempre accade, anche questa volta la maggioranza non ci ha ascoltato, non si confronta e non si mette in dubbio. Pertanto la situazione è ormai al limite.

continuiamo a credere che anche questa volta saremo costretti ad intervenire e che interverremo di nuovo con altri decreti-legge. Peraltro, uno studio recentemente pubblicato dalla Camera dei deputati ha evidenziato che a tutt'oggi

Forse è opportuno interrogarsi se con queste risorse si poteva fare altro, se si potevano spendere meglio, se si poteva mettere in campo una soluzione diversa.

Per tutte queste motivazioni, ma anche per altre, voteremo convintamente in Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel corso degli ultimi decenni si è registrata una profonda modifica strutturale del settore siderurgico, legata soprattutto alla globalizzazione della produzione, che ha generato una crisi che ha colpito soprattutto le grandi imprese. Non a caso il Parlamento è stato impegnato ultimamente nella risoluzione di problemi critici connessi alle nostre più grandi imprese del settore, l'ILVA *in primis*, ma anche la Lucchini, con gli impianti di Piombino Si tratta di realtà che si assomigliano sotto diversi aspetti e che hanno una matrice comune, quella della crisi economico-finanziaria, e che comunque sono riconducibili ad una carenza di politica industriale nel Paese, oltre che ad una mancanza di visione di insieme nel settore siderurgico nazionale. L'industria siderurgica italiana, al pari di altre realtà internazionali, non ha storicamente fruito di una volontà politica indirizzata a difendere e tutelare le eccellenze: ciò ha favorito la penetrazione nel settore di colossi internazionali, la cui missione è estranea alla tutela dell'eccellenza siderurgica e all'interesse del mantenimento della produzione italiana.

molto chiare neanche su quanti decreti-legge siano stati fatti per salvare l'ILVA. Sono stati capaci di nominare garanti, commissari straordinari, subcommissari, comitati di esperti, una squadra infinita di consulenti, ingegneri e tecnici, in anni di battaglie perse per questioni istituzionali e giudiziarie, anni di conflitti tra periti, giudici e ambientalisti, anni dove nulla o quasi nulla è cambiato, signora Presidente, anni che sono serviti solo ad aumentare la rassegnazione e la paura tra la popolazione tarantina. Noi consideriamo la storia dell'ILVA come qualcosa di drammatico, che impegna le Aule parlamentari dalla scorsa legislatura e che il Governo dei tecnici non ha saputo affrontare e risolvere con la dovuta concretezza. La vicenda dell'ILVA ha fatto soprattutto emergere tutta la fragilità del nostro sistema amministrativo di intervento nelle questioni ambientali e di politica industriale. La mancanza di chiarezza sui ruoli e sulle competenze degli organi istituzionali interessati al risanamento ambientale e alla riqualificazione del territorio di Taranto ha alimentato una serie di procedimenti penali e amministrativi con controbattute del Governo risultate fino ad oggi inefficaci,

soprattutto permesso l'intervento dell'autorità giudiziaria su questioni che rientrano chiaramente nella sfera delle competenze delle autorità garanti della tutela dell'ambiente e delle direttive comunitarie. Riteniamo che sia stata messa in gioco l'affidabilità e la credibilità del nostro Paese nei confronti degli investitori esteri. I cittadini di Taranto pagano l'irresponsabilità della classe imprenditoriale ed industriale del passato e l'irresponsabilità della classe amministrativa locale, che fino ad oggi ha chiuso ha chiuso gli occhi al problema sanitario e ambientale. I problemi ambientale e sanitario sono ancora più gravi se si pensa che nella stessa situazione di emergenza ambientale e sanitaria di Taranto ci sono anche altri cinquantasette siti di interesse nazionale, per la maggior parte situati al Nord del Paese, verso i quali il Governo deve intervenire con risposte concrete a tutela della salute dei cittadini. quattro anni dalle prime indagini della magistratura sul caso ILVA e sull'inquinamento dell'area di Taranto, abbiamo l'obbligo di guardare al passato soprattutto per capire e per tirare le somme sui risultati conseguiti nel percorso degli interventi tracciata dagli ultimi Governi. Questo è un atto dovuto nei confronti soprattutto dei lavoratori che hanno legato la propria vita e quella della loro famiglia al destino di quello che ancora oggi è il colosso siderurgico più importante d'Europa.

il loro futuro e come mantenere il lavoro. Se un'azione del Governo è sottoposta a così dure critiche da parte dei lavoratori, qualcosa sicuramente non va e non saranno certo dieci o undici decreti o undici decreti ad attenuare la loro rabbia. L'incertezza che ne deriva rischia di mettere in discussione l'attività dello stabilimento e far perdere commesse e affidabilità perché, al di là degli aspetti legislativi e burocratici e delle inchieste giudiziarie, vi è il lavoro quotidiano che va avanti grazie all'impegno dei lavoratori che, anche nei momenti più difficili della storia dello stabilimento siderurgico, si sono dati da fare

avete stoppato il dialogo; in Commissione in dieci minuti avete bocciato tutti gli emendamenti; avete avuto paura di confrontarvi in Assemblea; avete avuto la fretta di chi non accetta critiche e la discussione; avete avuto l'arroganza di pensare di avere voi e solo voi la verità in pugno. E forse, signora Presidente, anche la ministra Boschi si è un po' vergognata di venire in Aula a porre per l'ennesima volta la questione di fiducia.

Presidente, onorevoli colleghi, il passaggio parlamentare per la conversione in legge del decreto-legge n. 98 del 2016 fa seguito a quello di cui ci siamo occupati non più tardi di sei mesi fa, e questo è estremamente indicativo di quanto forte continui ad essere l'emergenza nel territorio sia per quanto riguarda le legittime preoccupazioni ambientali e di salute da parte dei cittadini, ma anche per quanto riguarda le refluenze lavorative, occupazionali e di politica economica che la questione comporta. Certamente la situazione del territorio ove insiste anche l'ILVA - e dove anch'io vivo e non a caso ho usato l'espressione «anche», perché le criticità ambientali presenti nel territorio di Taranto non vanno imputate esclusivamente alla presenza dell'ILVA, ma all'effetto cumulo derivante da diversi e importanti impianti inquinanti. Il fenomeno è presente in diverse città che ospitano poli industriali inquinanti, come Gela, Priolo, Gargallo, Augusta, Marghera o Ravenna. Potrei citare gli effetti della presenza delle raffinerie in questi poli. A Taranto la raffineria porta il nome di AGIP e anche a causa di tali presenze la qualità della vita della cittadinanza è diventata sempre più scadente, abituando fatalmente la gente a dover fare i conti con l'insorgenza di patologie la cui eziologia oggi è pacificamente messa in rapporto di causalità o concausalità con il degrado delle matrici ambientali aria, acqua, suolo. Malattie, quindi, ma anche esiti letali di queste malattie. Una situazione, quindi, che è peggiorata nel tempo e che tutti sappiamo non essere risolvibile in un batter d'occhio. Tuttavia si doveva pur iniziare, e non certamente per l'incombere della procedura di infrazione europea, ma perché è cosa giusta e necessaria per la sopravvivenza fisica ed economica di un territorio e dei suoi abitanti. E si è iniziato. Il Governo ha posto in essere delle azioni, ha individuato un percorso, ha sperimentato la necessità di aggiustamenti nel percorso, nella consapevolezza che quando si affrontano situazioni cosi complicate, non si è mai certi che il passo successivo sarà quello finale ed ultimo, risolutivo di ogni problema. si è fatto un passo in avanti nel raccogliere le manifestazioni di interesse relative all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali dell'ILVA. Sappiamo che hanno risposto 29 soggetti, di cui 17 italiani e 12 stranieri e che 19 di questi sono stati già ammessi alla fase di *due* *diligence*, e sappiamo come adesso si apra la fase nevralgica dell'individuazione di un soggetto solido e adeguato che possa garantire un futuro sereno al presidio industriale. Certo, ci muoviamo in un terreno delicato, in bilico sempre tra i vincoli europei che impongono il divieto degli aiuti di Stato alle aziende e la necessità di non dimenticare mai che cosa ha rappresentato l'ILVA per la siderurgia italiana, per il Mezzogiorno e per l'intera economia del Paese. E così, in discussione generale, abbiamo sentito le opposte valutazioni su quello che è forse l'aspetto più dibattuto dell'intero decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire, e cioè quanto contenuto all'articolo 1, comma 1, laddove si prevede che l'onere di restituzione dell'importo erogato dallo Stato ai sensi del precedente decreto n. 191 del 2015, per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo ILVA oggi 300 milioni di euro), sarà posto a carico dell'amministrazione straordinaria del gruppo e non più a carico dell'acquirente che si sarà aggiudicato la procedura di cessione. Abbiamo sentito quanti laceranti contrasti su questo e altri punti del decreto vi sono stati tra le formazioni politiche e ciò è sintomatico di come in Italia si sia ancora ben lontani dal conseguimento di un'unità nel concepire il rapporto con l'industria. Noi l'abbiamo già detto in passato e torniamo a ribadire che la siderurgia ha rappresentato e rappresenta ancora per il nostro Paese un settore strategico, ma è anche vero che il tema della sostenibilità ambientale, come anche del recupero ambientale dei territori degradati, deve essere un riferimento costante dell'agire di ogni amministratore e di ogni decisore politico, nel convincimento che un equilibrio è possibile e che un percorso di risanamento sia indispensabile. Rispetto a questo, e anche ILVA vi rientra pienamente, ci sono delle garanzie irrinunciabili e non negoziabili che devono essere realizzate: è fondamentale che gli stabilimenti non chiudano e venga quindi garantita la continuità operativa nel rispetto delle prescrizioni ambientali; bisogna garantire i livelli occupazionali e la sopravvivenza di migliaia di famiglie di lavoratori dello stabilimento e dell'indotto; bisogna garantire l'assoluta compatibilità ambientale delle produzioni; va garantita la tutela, soprattutto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto. Tutto questo comporta senso di responsabilità e questo senso di responsabilità noi del Gruppo AL-A vogliamo dimostrare, approvando il testo in esame e dando fiducia al percorso individuato per riallocare sul mercato i complessi aziendali e approdare al più presto all'auspicata stabilità industriale, finanziaria e gestionale. Non possiamo farci sedurre dal canto delle sirene che invocano improbabili retromarce. Anzi, partendo proprio dalla vicenda ILVA, il Parlamento deve rilanciare e focalizzare l'attenzione sull'attività di tanti altri

Pretendiamo il massimo coinvolgimento delle Commissioni competenti. Vigiliamo affinché quelle garanzie irrinunciabili di cui prima parlavo siano perfettamente rispettate. Esigiamo trasparenza e massima correttezza. Esigiamo responsabilità e senso del dovere. La storia di un Paese, di un grande Paese come il nostro, è fatta di passi concreti e di scelte lungimiranti che guardino al futuro e siano capaci di realizzarlo. Si può anche mettere in conto l'errore. Si può anche mettere in conto un difetto di valutazione, ma certamente non si può avallare l'immobilismo o, peggio, l'indifferenza. Il presente ci interroga ed esige da noi posizioni chiare e determinate. Noi siamo convinti che dobbiamo guardare alla storia di chi ha preceduto con gli occhi grati nei confronti di chi pensava di realizzare qualcosa di importante per le generazioni future, magari sottovalutando, a torto, che le risorse naturali fossero infinite o inesauribili. Oggi il presente ci chiede atteggiamenti più sensibili, valutazioni differenti, azioni più energiche nel considerare gli effetti cumulo degli impianti inquinanti che insistono in un medesimo territorio. Coniugare in maniera intelligente sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e della salute è una cosa possibile e la vicenda ILVA può e deve rappresentare per il nostro Paese un'esperienza un'esperienza di cui fare tesoro, ma anche una sfida per un cambio di rotta risoluto e serio che ponga al centro di tutte le decisione il benessere dei cittadini sotto ogni profilo ovviamente: sociale, economico, ambientale, sanitario; in una parola, il benessere umano. Interpellati da questo senso di responsabilità e motivati dalla necessità di non fermarsi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie.

il ricorso a un ulteriore decreto-legge a questo punto inevitabile per garantire il prosieguo dell'attività economica di un importante stabilimento a livello nazionale, direi ancor più internazionale, e al contempo provvedere a un risanamento ambientale serio, realisticamente possibile e definitivo, che le procedure esistenti non avrebbero potuto consentire.

Su una in particolare mi vorrei soffermare, e cioè in merito alla questione pregiudiziale - se non ricordo male - della collega De Petris, che richiamava supposti profili di incostituzionalità del decreto-legge. Devo rilevare che i relatori, e in particolare il senatore Orellana, si sono lungamente soffermati sui presunti criteri di incostituzionalità delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge in esame,

che già allora prevedevano la esclusione della responsabilità sia penale che amministrativa del commissario straordinario, che ora si è inteso estendere all'affittuario o acquirente,

Rispetto ai rilievi di costituzionalità la Corte ha, infatti, dichiarato inammissibili quelli riferiti agli articoli 25 e 27 della Costituzione e infondati tutti quelli riferiti agli altri articoli della Carta, tra cui in particolare l'articolo 3 più volte citato - forse in modo inopportuno - in quest'Aula. Un'ulteriore seconda e definitiva riflessione

delle questioni pregiudiziali - avrà il compito di valutare i piani ambientali presentati dai privati, come se si andasse a prefigurare una sorta di privatizzazione di una funzione che - come si sa - è tipicamente svolta dal Ministero dell'ambiente. bene ricordare che i tre esperti sono stati definiti in quanto aventi una competenza specifica e sono stati opportunamente nominati con decreto ministeriale. Ciò vuol significare che risulta infondata una sorta di accusa di privatizzazione di una funzione che è svolta dal Ministero e che è in capo al Ministero stesso.

esame viene ancora una volta imposto a quest'Aula con una richiesta di fiducia per la verità assolutamente accelerata, essendo

Il testo in esame rappresenta - a nostro avviso - proprio plasticamente la storia di un fallimento: un fallimento sotto l'aspetto industriale, un fallimento per la tutela della salute pubblica; un fallimento delle bonifiche e del risanamento di tutte le matrici ambientali e a pagarne le conseguenze sono soprattutto i lavoratori dell'ILVA, la loro sicurezza, i cittadini dell'area di Taranto per la crisi sanitaria e ambientale irrisolta e tutto l'ambiente circostante. Vorrei ricordare in questa sede che sono ancora al palo le opere di ambientalizzazione e di risanamento del territorio, così come tutte le misure di sorveglianza e tutela sanitaria. alcun risultato significativo sotto l'aspetto della riduzione dell'esposizione a inquinanti di origine industriale e dell'abbattimento dell'inquinamento. Sì, qualche lieve e saltuario segnale di miglioramento c'è stato, ma sapete perfettamente che è dovuto è dovuto solamente alla riduzione della produzione. Ciò significa che, in totale assenza di interventi ambientali strutturali, l'inquinamento atmosferico tornerà a salire e tutto ciò è inaccettabile per la salute dei cittadini di Taranto e per questo Paese. Insomma, ci troviamo di fronte a una perdurante e gravissima emergenza industriale, sanitaria e ambientale che ci si ostina ad affrontare con provvedimenti d'urgenza che, emanati praticamente senza soluzione di continuità, non hanno prodotto alcun miglioramento e non modificano l'attuale situazione. All'urgenza di interventi volti a ripristinare la qualità dell'ambiente e a dare soluzione alla drammatica situazione epidemiologica confermata in più occasioni nell'area di Taranto, il decreto-legge non trova di meglio che rispondere con la previsione di un'ennesima proroga, fino a un ulteriore anno e mezzo, per l'attuazione del piano ambientale e sanitario e con la possibilità di poterlo modificare secondo le esigenze, le convenienze dei futuri soggetti acquirenti. In pratica, vi è la riscrittura e la cancellazione delle prescrizioni, magari a cominciare proprio dalla copertura dei parchi minerari, che sarà proposta dai privati come condizione senza la quale l'acquisto non potrà avvenire. Quindi, se da una parte il provvedimento in esame è attento, molto attento, a favorire i nuovi acquirenti e ad agevolare la vendita dell'ILVA, prevedendo, tra l'altro, che non debbano essere loro a rimborsare i 300 milioni più interessi (quasi 400 milioni) erogati per esigenze finanziare del Gruppo, ma dovrà essere l'amministrazione straordinaria, quindi lo Stato; dall'altra il decreto-legge rimette di fatto in discussione lo stesso processo di ambientalizzazione dell'ILVA, così come previsto dall'AIA, che è presupposto per salvare lo stabilimento. Con ciò si fanno crescere e accrescere notevolmente le preoccupazioni di chi in quei territori vive e vive sulla propria pelle il disastro ambientale e sanitario. Dispiace

si prevede, infatti, che i futuri acquirenti o affittuari possano presentare proposte di modifica del piano ambientale e che tali proposte saranno valutate da un comitato di esperti. Vede, senatore Romano, noi crediamo proprio che l'ulteriore invenzione del comitato di esperti sia assolutamente incostituzionale. È evidente a tutti, infatti, che, mentre da una parte si continua a fare in modo che l'ARPA non possa avere l'organico sufficiente, dall'altra si istituisce detto comitato che riteniamo essere una vera e propria privatizzazione di una funzione svolta dal Ministero dell'ambiente,

su alcuna norma che eviti possibili conflitti di interesse tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici; nessuno - ad esempio - si può occupare ed è esperto in materia di epidemiologia e di tutela sanitaria. essere data priorità a quelle offerte di acquisto in grado di garantire una prospettiva di sviluppo vera, centrata sulla innovazione tecnologica e ambientale e sulla conferma degli attuali livelli occupazionali. Ma di tutto questo non vi è traccia nel provvedimento, così come non vi era traccia nei provvedimenti d'urgenza precedenti. Si interviene nella procedura riguardante le modifiche e le integrazioni al piano ambientale, definendo un'altra procedura nuova, secondo la quale il soggetto che presenterà un'offerta vincolante non solo potrà chiedere modifiche in relazione all'attuale piano ambientale e sanitario, ma anche ottenere il differimento, fino a diciotto mesi, del termine ultimo per l'attuazione delle prescrizioni previste. Il termine, che era già stato prorogato al 30 giugno 2017, diventa ora, ancora una volta, prorogabile di un anno e mezzo: una inaccettabile proroga di un termine già più volte differito, che si tradurrà in un ulteriore spostamento in avanti delle misure di risanamento ambientale previste dall'AIA e, quindi, delle opere di ambientalizzazione e di risanamento del territorio, senza imporre un preciso e vincolante cronoprogramma degli interventi di risanamento ambientale. È quindi una previsione - a nostro avviso - insostenibile, inaccettabile, anche perché l'attuazione delle misure previste dall'AIA rimane il presupposto essenziale per garantire la soluzione della gravissima emergenza sanitaria e ambientale.

fortuna approvato anche la legge sui reati ambientali. L'ulteriore ampliamento - conferma dello scudo precedente e ampliamento dello scudo attuale anche ai futuri

guardando esattamente e accettando una serie di emendamenti che noi abbiamo presentato, come hanno fatto altre forze politiche. Ma questo, come al solito, non è stato possibile. Per questo motivo, non solo non solo voteremo contro la fiducia, ma siamo assolutamente contrari nel merito a questo ennesimo decreto che rappresenta - e lo sosteniamo con forza - non soltanto la rappresentazione di un fallimento, ma una vera e propria regressione rispetto anche ai precedenti e

MPL))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, siamo alla conversione dell'ennesimo decreto ILVA, il decimo, e ancora una volta con una richiesta di fiducia. Quest'annosa vicenda riguarda un complesso aziendale che, per le sue dimensioni e per l'alto numero di dipendenti, è il più grande del nostro Paese ed è sicuramente quello che presenta un impatto ambientale tra i più significativi. Questo nuovo decreto riguarda il perfezionamento del precedente e mira alla soluzione di questioni relative alla cessione dei complessi aziendali, come disposto nel febbraio scorso. In altri termini, è utile - e non solo secondo me - a rendere più allettante la sua acquisizione da parte di una delle due cordate che sono in campo. Circa l'acquisto e la cessione dei complessi aziendali, voglio ricordare come fu gestita la prima cessione ai privati, quella del 1995, quando il dottor Emilio Riva poté subentrare in questa proprietà avendo a disposizione prepensionamenti di lavoratori anziani, da un lato, e contratti di formazione lavoro per l'assunzione di giovani operai, dall'altro. Si trattò di un'operazione praticamente a costo zero, anche per gli incentivi messi a disposizione. Non mi risulta che gli vennero chiesti, in quella occasione, impegni o investimenti per la sicurezza degli impianti, per il ciclo produttivo e sulle nuove tecnologie, né tantomeno per l'inquinamento. Con quella scelta gli fu offerta la licenza per inquinare e avvelenare un territorio, con il rischio che le persone si ammalassero e, molto spesso, morissero. Qualcuno parlò di una drammatica, tragica, regalia. Dopo l'epoca di Riva e il commissariamento sono state tantissime le promesse e gli impegni non mantenuti per affrontare e cercare di risolvere una situazione che si è fatta via via sempre più tragica, per la fabbrica, ma soprattutto per la città di Taranto e per il territorio circostante. Per ogni decreto d'urgenza approvato sull'ILVA ci è stato spiegato che si trattava di provvedimenti straordinari, in grado di arrivare all'esito di rendere esigibili i diritti costituzionali alla salute e al lavoro anche da parte dei cittadini di Taranto e dei dipendenti della fabbrica. Lo abbiamo fatto dieci volte in quattro anni (anzi undici, perché uno non era un decreto) fino ad approdare a quest'ultimo, che favorisce solamente la cessione ai privati. Il punto è che nulla cambierà con l'approvazione di questo decreto-legge al nostro esame ma, anzi, le misure che contiene peggioreranno la situazione attuale, dei cittadini e dei lavoratori. La fabbrica ha continuato a produrre gravi danni sulla popolazione e sull'ambiente. Con lo slittamento di diciotto mesi del termine di attuazione del piano di tutela ambientale e della salute approvato dal Consiglio dei ministri nel marzo 2014, prevediamo un ulteriore allungamento di tempi per un piano che era già stato licenziato in ritardo ed era già intervenuto spostando in avanti l'applicazione delle prescrizioni dell'autorizzazione territorio e del mare dichiarò che questo sarebbe stato lo strumento per risolvere i drammi di Taranto e che, subito dopo, il commissario straordinario avrebbe predisposto il piano industriale. Ma quale piano industriale! Il commissario aveva questo compito, ma non è riuscito a svolgerlo (non si trattava neppure di un compito che gli era proprio, in quanto demandato dal Governo). Nessun risanamento è stato fatto - zero

sono stati spostati ulteriormente in avanti (fino al giugno 2017) per arrivare, ad oggi, a una norma che consente a chi presenterà un'offerta vincolante di richiedere modifiche al piano ambientale e un differimento fino a diciotto mesi del suo termine ultimo.

Ma c'è di più. Parliamo infatti dell'estensione dello scudo giudiziario già previsto per i commissari anche ai futuri acquirenti e affittuari e ai loro delegati. Questa norma consentirà loro di non rispondere penalmente, civilmente e dal punto di vista amministrativo delle condotte che porranno in essere.

Solo in questo modo ci sarebbe stata una certezza per i lavoratori. Si profilano giornate dure per tutti gli operai, che sono circa 12.000.

ormai incondivisibile, che tende a non creare discontinuità con un passato insostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Si abbia il coraggio di dire che l'industrializzazione inquinante in territori come Taranto (ma potrei citare altri poli industriali come Ravenna, Gela o Augusta) ha fatto il suo tempo e che ora è necessario puntare alla riconversione delle aziende che, come priorità assoluta, devono perseguire la compatibilità totale con l'ambiente. Altro che slittamento dei piani ambientali!

È inutile agitare lo spauracchio della perdita dei posti di lavoro o del detrimento per l'economia nazionale, se questo è il prezzo da pagare. Ci sono valori e beni non negoziabili e la salute dell'uomo e dell'ambiente è tra questi. È passato tanto tempo, fin troppo, e non ci sentiamo di condividere ulteriori strategie del ritardo, tantomeno se condotte sotto la mannaia della questione di fiducia. è per questi motivi che, che pur nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Gruppo cui appartengo, annuncio il voto contrario del Gruppo Grandi Autonomie e

è, già di per sé, assolutamente anomalo. I contenuti del decreto-legge sono stati ampiamente illustrati in discussione generale. Il decreto sinteticamente riguarda la questione delle procedure di cessione a terzi, affronta i diritti essenziali della tutela della salute, della tutela dell'ambiente e della tutela del lavoro. Cura, tra l'altro, con particolare attenzione la questione della restituzione degli importi erogati e, quindi, in un certo qual modo, avvia e rafforza quelle procedure che sono tendenti all'affidamento a terzi dello strategico impianto sotto forma di forma di vendita, di affitto o di cessione di altra natura. L'obiettivo fondamentale nell'interesse del Paese credo sia quello di avviare una seria riconversione e rimodernizzazione degli impianti, curando evidentemente in maniera particolare i principi della tutela della salute e dell'ambiente e, ovviamente, la salvaguardia e le garanzie occupazionali che devono riguardare non soltanto gli occupati dell'ILVA, ma anche di tutte le aziende che lavorano nell'indotto. Questo è in spiccioli il contenuto sostanziale del decreto-legge.

è arrivata ad un punto di non ritorno e, quindi, evidentemente, bisogna continuare ad affrontarla e gestirla proprio perché un complesso così grande, il più grande complesso siderurgico d'Italia, il

la politica e il Parlamento non si sono mai interrogati e non si sono mai dati una risposta compiuta sulla questione ambientale di Taranto; una questione ambientale che non è ascrivibile esclusivamente o principalmente agli impianti dell'ILVA e, devo

Quindi, evidentemente, si partiva già da una situazione ambientale e gestionale gravemente compromessa.

ma riguarda anche lo Stato italiano perché, prima o poi, ci dobbiamo interrogare sulla gestione del bacino militare, gestito dalla Marina militare; ci dobbiamo interrogare prima o poi anche sulla gestione di quella cantieristica militare e, quindi, di quella attività di ricovero e demolizione

Non possiamo poi sottacere anche una nostra nota critica perché evidentemente, pur nella positività di questo decreto-legge che andremo a votare,

e, in particolare, l'ultima erogazione da 300 milioni potrebbe anche non essere restituita e quindi potrebbe anche gravare definitivamente sulle casse dell'erario, senza sciogliere i nodi dell'aiuto di Stato.

deve pagare l'inquinamento e il disastro ambientale prodotti nell'arco di questi decenni in quel sito industriale? Chi dovrà affrontare tale questione se, come dicevo prima, il disastro ambientale

perché c'è la reale perplessità che un'insolvenza dell'azienda possa mettere a repentaglio la restituzione dei 300 milioni.

Se, da un lato, ci convince l'idea che, di fronte ad una situazione straordinaria, possa essere assunta una decisione straordinaria, ovvero quella di conferire un livello di immunità penale a chi dovrà gestire per i primi tempi l'impianto, andando in deroga

per quale periodo, per quante persone e per chi vada esteso questo criterio dell'immunità. Riguarderà soltanto l'acquirente, solo l'amministratore delegato

altre ne sono state introdotte. Mi riferisco a un emendamento, inserito in sede di conversione alla Camera dei deputati, che pone un'attività di monitoraggio e di mappatura dei rifiuti pericolosi e radioattivi e radioattivi in capo alla gestione commissariale senza affrontare la questione della relativa copertura finanziaria. Da questo punto di vista abbiamo anche delle perplessità sulla legittimità di questo decreto-legge che almeno per questo profilo specifico, potrebbe essere privo della debita

perché, nel calcolo del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, ci rendiamo conto che è necessario continuare sulla strada che il Parlamento e i Governi che si sono susseguiti hanno intrapreso da tempo. Facendo parte di una maggioranza, ci rendiamo conto che, talvolta,

l'equivalente dello stipendio di solidarietà di un operaio dell'ILVA. Tutto ciò che un operaio avrà dato in undici mesi verrà bruciato in soli dieci minuti. La follia di un tale progetto, chiamato ILVA di Taranto, risiede in questi numeri, che possono essere allargati: diventano 2,5 milioni al giorno - basta fare una semplice moltiplicazione - oppure circa 1.090 milioni all'anno. Per dirne un'altra, negli ultimi quattro anni l'ILVA ha perso 3 miliardi e 90 milioni di euro. Anche il mito per cui l'ILVA sarebbe una società competitiva a livello nazionale e internazionale è dunque falso. Chi dovrebbe mettere i 3 miliardi di euro? Li dovrebbe mettere chi se la compra,

evidenziare: nel momento in cui si stabilisce che la contaminazione è certa, ci si trova nella situazione per cui i lavoratori lavorano in condizioni di accertato pericolo. Ipotizziamo che ci sia una contaminazione diffusa da amianto e da residui radioattivi o da diossina: in teoria vanno forniti ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale atti a cancellare il rischio di contaminazione o di morte. Questo è quanto dovrebbe venire fatto. Pensate che si faranno lavorare 10.000 persone in queste condizioni o troveremo una deroga? un'altra cosa bella: avete scritto che chi compra non è responsabile dell'inquinamento pregresso. Suonerebbe anche bene: quindi non paga chi compra. E gli altri? I Riva non pagano perché non hanno i soldi. Quindi, chi paga

Analizziamo la procedura con cui intendete andare avanti. Prima di tutto, il termine per realizzare il piano degli interventi ambientali e sanitari viene spinto in avanti, e questo è un Gli eventuali acquirenti - cioè gli interessati all'acquisto - avranno la facoltà di proporre un'alternativa, cioè di rinegoziare l'AIA come vogliono loro. Poi, un comitato di esperti avrà centoventi giorni per esaminare e intanto vengono buttati via Al termine di questo passaggio si comunicheranno agli eventuali acquirenti i risultati dell'analisi delle loro proposte. Gli acquirenti avranno modo di dire sì o no: a un certo punto, uno o più potenziali acquirenti diranno sì e faranno un'offerta vincolante. A quel punto

per le misure di tutela ambientale e sanitaria. Ebbene, di questi 530 milioni di euro, 860.500 euro sono stati spesi per quello ben 529 milioni di euro su 530 sono stati spesi per altro. La morale è che sono stati spesi per pagare i fornitori o, eventualmente, per adeguamenti impiantistici. Quindi, chi viene a raccontare che l'Unione europea non potrà dire nulla o non è chiusa ancora la procedura di infrazione sta solo allungando i tempi, perché di fatto il decreto-legge ILVA al nostro comprando tempo, facendolo pagare ai cittadini italiani. Questo è quanto state facendo. Ma prima o poi la realtà vi raggiungerà, anzi vi supererà, e ci sbatterete la faccia contro. Questo succederà. Parliamo ora dei 300 milioni. Prima li avrebbe dovuti restituire chi avesse comprato l'ILVA; adesso li deve restituire l'amministrazione straordinaria, che non è un soggetto giuridico, non è una srl, non è una snc, non è una società per azioni. Non è niente; però ha contratto un debito con lo Stato di 300 milioni e li ha spesi, quindi non può restituirli, perché i commissari non sono né civilmente, né penalmente responsabili. Quindi non posso portarli in tribunale e chiedere loro conto dei 300 milioni. milioni. Sapete come si chiama? Si chiama *bad company*. Voi avete creato una società fittizia, che non esiste giuridicamente, che è responsabile di quei 300 milioni e che non li potrà mai restituire. Il cittadino italiano ringrazia sentitamente.

anzi, questo no andava detto prima. Però mi meraviglio che voi vi lamentiate di questo. Voi continuate, con la vostra riforma costituzionale, a dire che bisogna cambiare per fare le riforme economiche. Bene, il vostro cambiamento su questo argomento è diventato la reazione più pura. Non siete conservatori: siete reazionari, siete restauratori, aggrappati a un dinosauro. Questo siete. M5S).* Avete parlato della necessità di una Costituzione diversa per fare una riforma economica, ad esempio una pianificazione industriale. E allora fatela. La potevate fare con questo decreto, senza bisogno di cambiare la Costituzione, però non l'avete fatto. Ciò vuol dire che anche il cambio costituzionale è solo un pretesto, fumo negli occhi dei cittadini, ma anche vostri, naturalmente, che mangiate pane e fumo, come fu detto dalla mia collega Elena Fattori in un altro momento. Evidentemente vi piace il fumo senza l'arrosto. Vorrei dire un'altra cosa. Quando vi riempite la bocca di Taranto e dei lavoratori, ricordatevi questo: l'ILVA, è vero, ha prodotto acciaio, che è diventato in parte acciaio inossidabile e che ha riempito tutta l'Italia. Quando cucinate la pasta e usate una pentola di acciaio inossidabile fatta con l'acciaio dell'ILVA, ricordatevi che quella roba lì gronda sangue. Voi state mangiando con pentole rosse di sangue e con posate rosse di sangue: il sangue della gente di Taranto. A Taranto ci sono 200.000 persone che subiscono gli effetti di quello che voi fate qua, per salvare 11.000 posti di lavoro. Ma se il vostro problema sono queste 11.000 persone, con gli ammortizzatori sociali spendereste sicuramente di meno. È una questione di visione futura e invece voi state aggrappati al passato. Quanto costa mantenere questi posti di lavoro, in termini sanitari e ambientali? Chi se ne frega, naturalmente. Ma andiamo avanti. Cosa proponiamo noi per il futuro, visto che quello è il passato e bisognerebbe solo dimenticarlo? Voi vi riempite la bocca con il fatto che bisogna fare ricerca e innovazione. Bene, la produzione di massa di acciaio è una cosa che nell'Europa occidentale non ha più senso. Non abbiamo più questa necessità di costruire, costruire e costruire; ce l'ha la Cina e ce l'ha l'India, ma non ce l'abbiamo noi. Ecco perché la produzione cinese è ultracompetitiva rispetto alla nostra. L'ILVA è fuori mercato da qualunque punto di vista: non può produrre utili e non potrà farlo mai più,

Quindi, dato che questa è una cosa fuori mercato, bisogna pensare a qualcosa che ha senso adesso e che non ce l'aveva prima: si chiama economia di scala. I grandi siderurgici servivano per avere un'economia di scala nella produzione. Adesso esiste una cosa che si chiama manifattura additiva che permette di produrre dei pezzi industriali in modo impossibile in altra forma: pezzi aeronautici, dove la tecnologia è al massimo. Bene, una delle idee che abbiamo noi, una volta lavorato per cent'anni per smantellare quello che c'è, è di fare un bel distretto della manifattura digitale. Un'altra cosa di cui c'è bisogno in quella zona è un programma di disinquinamento. Noi siamo all'avanguardia per il *decommissioning* nucleare; possiamo diventare all'avanguardia anche per il *decommissioning* chimico. Questo è pensare al futuro; invece voi pensate al passato. Chiudo dicendo un'ultima cosa. Ho guardato i dati occupazionali: nel tarantino la disoccupazione è cresciuta negli ultimi cinque anni e, sommata al tasso di inoccupati, si arriva al 47 per cento. Quindi l'ILVA non ha risolto e non risolverà mai i problemi occupazionali di quella zona. Quindi è ora di voltare pagina, basta con il passato. Voi siete dei dinosauri, e i dinosauri si sono estinti; dovrete estinguervi anche voi. Signora Presidente, colleghi senatori,

Parliamo di un'impresa con una storia ultradecennale, di un'importante realtà del nostro Paese che vanta tutti i suoi siti produttivi solo nel nostro territorio e che dà lavoro a quasi 15.000 connazionali, di cui ben 12.000 nel sito di Taranto. Parliamo di un'impresa che lo stesso Governo ha giustamente definito di «interesse strategico nazionale», in considerazione del ruolo chiave che riveste non solo per la siderurgia, ma anche per l'intera economia italiana. Parliamo di un'azienda che è il simbolo della nostra eccellenza nel mondo tanto da essere, addirittura, il il più grande sito produttivo d'Europa nel suo settore. Eppure sull'ILVA si continua, decreto dopo decreto, a procedere in maniera confusa e inadeguata, determinando così gravi ricadute sia in termini occupazionali che economici per l'azienda stessa, per le imprese del suo indotto e per la nostra economia. Questo provvedimento riconferma lo stesso modo di operare del passato, ed infatti emergono chiaramente vari aspetti che lo rendono inaccettabile. Il primo di questi è la sua incostituzionalità, sia per la scelta della decretazione d'urgenza che per la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Infatti, come ampiamente descritto ieri dalla questione pregiudiziale presentata da Forza Italia, il provvedimento è completamente privo dei requisiti di necessità ed urgenza indispensabili per l'utilizzo di questo strumento legislativo. È infatti solo Palazzo Chigi che vuole confronti muscolari con il Parlamento per privarlo delle sue prerogative costituzionali e imbavagliarlo con l'ennesima fiducia. Proprio il numero di fiducie costituisce uno dei due *record* di cui questo Governo si può fregiare; l'altro è il debito pubblico.

quarantacinque richieste dall'ultimo Governo Berlusconi, ma in un lasso temporale di tre anni e non di due, come ha fatto l'attuale Governo. Altro motivo che rende inammissibile questo decreto è la decisione di concedere la piena impunibilità oltre che all'amministratore straordinario, anche all'acquirente e ai suoi delegati, ponendoli così al di sopra degli altri cittadini, in pieno contrasto con l'articolo 3 della Carta costituzionale che sancisce, invece, l'uguaglianza dinanzi alla legge. Proprio questa estensione dello scudo giuridico, infatti, determina una zona d'ombra del diritto, in cui si inibisce il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale causando una profonda indeterminatezza su quali siano i limiti e soprattutto le responsabilità dei soggetti. Un pericolosissimo precedente in materia penale, soprattutto per un Paese come il nostro, che vede proprio nell'incertezza del diritto uno dei maggiori problemi di competitività delle nostre imprese nei confronti di quelle degli altri Stati. Il fatto che si voglia insistere sull'ampliamento dei beneficiari di questa impunibilità fa sorgere il dubbio che tale norma serva, come al solito, per proteggere «gli amici degli amici», al fine di coprire l'incapacità dell'attuale amministrazione straordinaria o, peggio, la gestione dei futuri acquirenti. E quindi, come diceva il grande statista e noto ex componente di quest'Assemblea: «A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca». Un ulteriore motivo per cui questo provvedimento è inaccettabile deriva dalla totale indifferenza del Governo verso le famiglie e il territorio di Taranto. Prevedere una proroga di 18 mesi del termine per l'attuazione del Piano ambientale e di risanamento dell'ILVA e di ogni altro adempimento ad esso connesso, rispetto alla precedente scadenza prevista per giugno 2017, rappresenta uno schiaffo a chi da anni è tormentato dai problemi sanitari e ambientali e che dovrà attendere fino al 2019 per avere tutela della propria salute. Inoltre, trovo inspiegabile che, in tempi di *spending review*, si possa autorizzare ARPA Puglia ad assumere personale a tempo indeterminato per la copertura delle future «attività di vigilanza, controllo, monitoraggio», duplicando così funzioni attualmente già in capo a ISPRA. Allo stesso modo, non pochi dubbi solleva la clausola che coinvolge la Cassa dei servizi energetici ambientali quale copertura degli oneri derivanti dai 400 milioni versati a favore dell'amministrazione straordinaria nel 2016. Una norma che, secondo le dichiarazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, gas e servizi idrici, potrebbe causare rincari in bolletta per i cittadini italiani. È proprio vero che la storia è fatta di corsi e ricorsi e la sinistra lo sa bene. Esattamente come Prodi, poco più di vent'anni fa, attraverso l'IRI, aveva messo in liquidazione l'allora Italsider, oggi la

Alla luce di quanto descritto finora, non si può che constatare che questo Esecutivo preferisce la comunicazione ad effetto agli effetti concreti che un buon provvedimento avrebbe potuto portare. Ma dopotutto, questo è il Governo delle false riforma che abolisce senza mai abolire, come fatto con Province e Senato, che governa senza aver chiesto il consenso dei cittadini, infatti non è passato da una consultazione popolare, che lancia proclami ma non fa i fatti, perché continua a procrastinare le decisioni. Insomma, mi pare proprio che l'Esecutivo si comporti come il Tancredi del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, che voleva cambiare tutto affinché nulla cambiasse. Ma purtroppo non siamo all'interno di un romanzo: il Paese, i cittadini e la nostra economia hanno bisogno di interventi reali per potersi riprendere e non bastano gli «zero virgola» per perseguire quella crescita di cui abbiamo bisogno. Questo non è il Governo che gli italiani meritano e sicuramente non è il Governo che hanno scelto ed è per questo che sono sicuro che al prossimo *referendum* i cittadini esprimeranno un secco e convinto no alle false riforme e alle false promesse dell'Esecutivo. Lo stesso no, per le motivazioni esposte, esprimiamo noi di Forza Italia a questa ennesima ed ingiustificata richiesta di fiducia su un provvedimento che non è stato certamente varato nell'interesse dei cittadini italiani e nell'interesse del Paese intero.

anche in questa occasione, tornando a discutere della vicenda ILVA, l'attenzione di tanti colleghi è stata attratta più dallo stucchevole dibattito sulla contabilità dei decreti-legge emanati nel corso di questi ultimi anni che dal futuro di quella realtà industriale e dalla complessità delle questioni che ad essa sono collegate. In realtà, proprio la ripetuta iniziativa legislativa cui si è fatto ricorso dopo l'intervento della magistratura di quel 26 luglio 2012 (proprio ieri quattro anni fa) semmai la conferma che siamo di fronte a quella che è, a mio parere, la più grave crisi industriale ed ambientale oggi aperta in tutta Europa e, nel contempo, al destino di ben 15.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti e del principale impianto siderurgico d'Europa dove si produce un terzo del fabbisogno nazionale di acciaio. Perché di questo stiamo parlando, non certo di una vicenda ordinaria. In questo dibattito, in cui non sono mancati i cedimenti alla retorica inconcludente e alla demagogia a piene mani, cui - devo dirlo - i colleghi Cinque stelle hanno mostrato anche in questa Aula, in queste ore, una qualche predisposizione, noi rivendichiamo con forza e coerenza lo sforzo, certo non privo anche di errori e approssimazioni, compiuto in questi anni: uno sforzo volto a tenere insieme - ripeto: a tenere insieme - l'emergenza ambientale e sociale di un'intera città con la necessità di salvare e valorizzare un pezzo decisivo del nostro sistema manifatturiero, a cui l'Italia non può e non deve rinunciare. Abbiamo scelto la strada che sapevamo essere la più difficile ed ambiziosa insieme. Altri hanno invocato, anche in questa occasione, scorciatoie e semplificazioni, utili solo a brandire la bandiera di una delle parti di questa così complessa vicenda, alimentando colpevolmente una rinnovata quanto anacronistica dicotomia tra ambiente e industria, tra salute e lavoro, che l'Italia e la stessa Taranto hanno più volte mostrato di voler superare. Vorrei invitare un attimo costoro e tutti noi a riflettere su quale sarebbe oggi lo scenario se Governo e Parlamento non fossero intervenuti: un complesso aziendale sequestrato e fermo, molte migliaia di lavoratori alle prese con gli ammortizzatori sociali e privi di qualsiasi futuro di stabile rioccupazione e la prospettiva dello stesso risanamento ambientale del sito industriale resa sostanzialmente impraticabile dall'assenza di risorse e dal venir meno di ogni legame con la continuità produttiva e aziendale. La realtà, invece e per fortuna, è che tale scenario è stato scongiurato in questi anni anche grazie agli interventi oggetto dei vari decreti-legge oggi a Taranto e per l'ILVA si aprono prospettive ben diverse, per quanto non ancora soddisfacenti, rispetto alla narrazione che i Gruppi di opposizione hanno voluto raccontare. alcuni fatti. Il piano ambientale approvato nel 2014 è in via di realizzazione, tant'è che sono state completate 112 prescrizioni e altre 58 sono in corso di attuazione, anche grazie alle risorse anticipate dal Governo, come è stato richiamato ieri sera dal collega Mirabelli. È stata assicurata la ripresa produttiva dello stabilimento di Taranto che è tornato a produrre tra i 5 e i 6 milioni di tonnellate annue. Non un solo lavoratore è stato licenziato anche grazie all'utilizzo sapiente e a turno degli ammortizzatori sociali. È stato avviato un piano graduale di pagamenti dei crediti all'indotto, mentre per le attività in corso vengono garantiti pagamenti regolari. Gli stessi interventi ambientali stanno dando i primi risultati: la città di Taranto è protagonista del primo Contratto istituzionale di sviluppo, a cui sono stati destinati circa 800 milioni di euro di risorse pubbliche per gli interventi di infrastrutturazione e bonifica della città e del porto. Mentre parliamo è in corso, a Palazzo Chigi, l'ennesimo incontro per il futuro dei 520 lavoratori del *terminal container* di Taranto. L'azione del commissario straordinario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione di Taranto - parliamo degli interventi rivolti alla città - sta producendo risultati importanti: sono stati ultimati i lavori relativi alla scuola Deledda del rione Tamburi e sono in corso di ultimazione i lavori di riqualificazione delle altre quattro scuole di quel quartiere; sono in corso i lavori relativi alle aree portuali e sono state completate le attività di caratterizzazione e di analisi dei rischi in molte aree della città e del Mar Piccolo. È stata avviata la messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi nel deposito ex Cemerad. Infine, è accaduto quello che probabilmente in molti auspicavano non accadesse mai: si sono costituite due cordate di importanti imprese e soggetti finanziari, che hanno presentato istanza per rendere contendibile la futura ILVA. Ciò ha visto la presenza anche di grandi aziende internazionali, che stanno partecipando alla procedura di acquisto smentendo in tal modo le cassandre che ritenevano che questo momento non sarebbe mai arrivato. Siamo ancora lontani dagli obiettivi che ci siamo prefissi, ma è falso e non onesto sostenere che in questi anni non sia accaduto nulla o che la situazione a Taranto e all'ILVA sia la stessa di quattro anni fa. lo stesso decreto-legge che ci accingiamo a convertire contiene misure che si iscrivono coerentemente nello sforzo profuso sin dall'inizio, a cominciare dalle modifiche che legano indissolubilmente e sempre più strettamente il piano industriale al piano ambientale e che costituiscono una maggiore tutela nei confronti degli *standard* di rispetto ambientale e di applicazione delle

da personalità del tutto autorevoli per competenza ed indipendenza e dal più esplicito coinvolgimento delle agenzie ambientali pubbliche. Particolarmente significativa, a questo proposito, è la norma approvata alla Camera con cui si autorizza l'ARPA Puglia ad assumere personale a tempo indeterminato per assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti proprio l'attuazione del piano ambientale. Ulteriori misure, come puntualmente richiamato dai relatori nella loro illustrazione, sono relative a meglio chiarire, peraltro in linea con le stesse indicazioni della Commissione europea, le modalità di erogazione e di rimborso delle risorse anticipate dallo Stato e destinate, in parte, a garantire la continuità produttiva ed occupazionale (300 milioni) ed, in parte (800 milioni), totalmente vincolate a finanziare gli interventi ambientali: risorse, queste ultime, su cui lo Stato potrà rivalersi in nome del principio per cui chi inquina paga. A proposito di queste risorse, è indicativo della strumentalità di alcune posizioni, ribadite anche in quest'Aula, il succedersi di interpretazioni le più varie e contraddittore. Abbiamo ascoltato varie tesi del tipo: siamo in presenza di regalie ai privati che acquisteranno l'ILVA (come se ciò dovesse avvenire *gratis*), lo Stato non ha messo alcun soldo sul risanamento ambientale (e abbiamo visto che è falso);

si tratta risorse anticipate dallo Stato con finalità ben chiare, che rientreranno nelle casse pubbliche in modo assolutamente lineare e per nulla aleatorio. ho avuto la possibilità di seguire da vicino in questi anni il percorso parlamentare dei vari interventi legislativi e il dibattito che li ha accompagnati in queste Aule e nel Paese. Ho grande rispetto per le opinioni diverse dalle nostre sulla bontà di questo come di altri provvedimenti, purché abbiano però l'intelligenza e, se posso dirlo, l'umiltà di cimentarsi con il merito delle misure adottate di volta in volta e con la complessità e la drammaticità della vicenda. Continuo a trovare, invece, alcuni toni ed argomenti francamente incommentabili per la demagogia e il velleitario benaltrismo, se così posso definirlo, privi di una qualsiasi proposta alternativa credibile a quanto fatto finora e di ciò non possiamo che prendere atto: evidentemente non si vuole cogliere la complessità della sfida che abbiamo dinanzi a noi. L'esito di questa sfida sarà decisivo, non solo per Taranto

un Paese che ha scelto da tempo di provare a declinare una moderna politica industriale fondata sulla sostenibilità dei processi produttivi e sulla piena coerenza con gli obiettivi di rispetto della salute e dell'ambiente. ILVA può e deve essere il battistrada di una nuova siderurgia tecnologicamente e ambientalmente all'avanguardia sul mercato globale. In questi anni, e ancora con questo decreto, ci ha ispirati sempre una caparbia volontà, politica ed istituzionale, di tenere insieme tali obiettivi e, in particolare, la continuità produttiva con il risanamento ambientale: non riconoscerlo, prima ancora che non onesto, è un errore madornale. Per tali ragioni, con altrettanta determinazione, continueremo a lavorare incessantemente per il futuro dell'industria italiana e per il bene dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e, proprio per avvicinare quanto più possibile questo futuro, i senatori del Partito Democratico voteranno con convinzione a favore della conversione in legge di questo decreto-legge e rinnoveranno la fiducia al Governo.

non vi nascondo una forma di disagio collegata direttamente al fatto che ci troviamo a votare l'ennesimo decreto salva ILVA, un provvedimento che ripercorre strade e soluzioni purtroppo già viste. Il mio giudizio su questo decreto-legge è scettico e sospettoso sull'impostazione, che non getta le basi per opzioni industriali credibili e sostenibili, sia economicamente che ecologicamente, in campo siderurgico. Per analogia di materia, essendo di Trieste e occupandomi attivamente delle problematiche della Ferriera di Servola del Gruppo Arvedi, ho seguito da vicino la vicenda dell'impianto siderurgico tarantino dove, nonostante i tentativi, non si è tuttavia riusciti a risolvere le conflittualità ambientali, sanitarie e lavorative esistenti tra la realtà industriale e la popolazione coinvolta. Credo che per quanto riguarda la città di Taranto - ma lo posso dimostrare anche nel caso di Trieste - gli indicatori di salute e di qualità della vita non lascino alcun dubbio. L'ILVA ci pone di fronte un tema che qualche volta tendiamo ad ignorare. *(Brusio).* PRESIDENTE. Scusi, senatore Battista. Pregherei di abbassare il tono delle conversazioni per consentire di ascoltare. Non riesco a percepire le parole del senatore Battista. Prego, senatore. all'obbligo di contemperare il diritto alla tutela della salute umana e ambientale con quello del diritto al lavoro e con la libertà d'impresa. Ciò che chiedo oggi a quest'Assemblea è, sì, creare le condizioni per fare impresa e risanamento ambientale ma, al contempo, riconoscere e valutare, all'interno di questa bilancia, i risultati in campo sanitario e di qualità della vita per gli abitanti tarantini, *in primis* per quelli che risiedono nel quartiere Tamburi. Sappiamo bene che il settore siderurgico europeo è da tempo in crisi e ha bisogno di essere ripensato, ben più profondamente di quanto ha fatto il piano Tajani per la siderurgia. In questo contesto, la situazione dell'ILVA spicca per la sua unicità. Per questi motivi, credo che la conversione del presente decreto-legge, come tutti gli interventi emergenziali, non sia che una soluzione incompleta, anche se necessaria, per una politica industriale più complessa che mi auguro trovi presto una soluzione definitiva. Anzi, per questo motivo chiedo al Governo di aprire un confronto di merito, che ci veda impegnati nell'esaminare proposte che modifichino o favoriscano una riconversione ecosostenibile e un reale ammodernamento delle strutture industriali esistenti, facendo facendo esperienza dell'innovazione tecnologica e industriale in chiave di sostenibilità economica e strategica per il Paese. Occorrono soluzioni che non pregiudichino posti di lavoro, non danneggino la salute delle persone e contribuiscano, per quanto possibile nella situazione attuale,

con 12 milioni di lire (quello era il valore della prima ILVA) è iniziata tutta una catena di aiuti di Stato. Mi riferisco, ad esempio, a quando

già stati fatti. Diciamo subito che nel 1995 i valori di emissione non erano adeguati neanche

diossine non sono cancerogene. Quindi, gli effetti sono ascrivibili fondamentalmente agli IPA, ai fumi di cokeria, ma questi venivano dagli altiforni precedenti. Premesso questo, dobbiamo

Ho sentito discorsi raccapriccianti: non è che se compriamo l'acciaio che arriva con le navi inquiniamo meno. Facciamo un discorso più globale, andiamo nel dettaglio delle questioni: quando gli IPA ricadono, a temperatura ambiente, sono liquidi; le polveri di ferro possono sporcare ed essere brutte da vedere, ma sono pesanti, cadono, non si respirano e non sono cancerogene. Cosa vuol dire? Che bisogna fare un investimento importante,

bene e di far male e quando c'è questa possibilità, è nella responsabilità di tutti fare le cose nel modo più trasparente e razionale possibile, ma questo non si fa a suon di titoli populistici sui giornali, che lanciano allarmi quando non c'è fondamento, si fa sulla base di dati

non parteciperà al voto in coerenza con la posizione storica e politica del Movimento associativo italiani all'estero, che non condivide l'abuso che questo Governo fa del ricorso allo strumento della la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.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

Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi,

Napolitano,

Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci,

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

interprete della necessità di tutelare i prodotti a denominazione di origine controllata, a denominazione di

delega all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la possibilità di produrre e installare quelle tecnologie elettroniche in grado di garantire i consumatori.

Presidente, all'articolo 5 abbiamo presentato diversi emendamenti e altrettanti ordini del giorno;

e di tutela della filiera agroalimentare rispetto alle posizioni dell'Unione europea.

Nel caso specifico, con l'ordine del giorno G5.100 si impegna il Governo «a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza». Signor Presidente, io vorrei che su questo punto vi fosse una seria riflessione da parte del Governo, non solo, come è proposto nell'ordine del giorno, a valutare che l'indicazione sia obbligatoria, ma ad impegnarsi affinché si apra un serio tavolo di confronto in sede europea e in maniera definitiva si giunga a mettere la parola fine a questa differenziazione per cui, alla fine, vengono tutelati i prodotti non definiti nella loro matrice italiana ma nella loro matrice commerciale. Mi spiego meglio. A noi interessa (e con questo ordine del giorno lo si specifica bene) che ciò che viene prodotto in Italia sia indicato come prodotto in Italia, che l'ingrediente principale sia indicato in maniera chiara e netta. Infatti, troppe volte ritroviamo con prodotti che danno l'idea di essere prodotti in Italia ma, nella realtà, contengono degli ingredienti primari provenienti da altri Paesi. Se ha un senso la tutela della filiera agroalimentare, questo non può essere confuso con il commercio.

giorno G5.101 si impegna il Governo a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari, al fine di tutelare il consumatore e la sua salute. Occorre fare attenzione, perché non possiamo dimenticarci che l'agricoltura ha delle necessità

ordini del giorno

parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 4

ha partecipato ai lavori della XIV, XV e XVI legislatura. Altri colleghi sono venuti a conoscenza della triste notizia e, forse, meglio di me avrebbero potuto parlare in quest'Assemblea circa la presenza del senatore Delogu nelle legislature che hanno preceduto l'attuale. Tra questi c'è Maurizio Gasparri che, con me, ha condiviso il cordoglio per questa notizia che, peraltro, era un militante, come il senatore Delogu, del partito di Alleanza Nazionale.

È stato anche molto apprezzato per la sua appartenenza al mondo sportivo. Egli è stato Presidente della società Cagliari calcio, è stato anche consigliere della Federazione italiana giuoco calcio per tantissimi anni ed è stato nel Gran giurì della UEFA. È dunque una persona che, anche nel mondo dello sport, ha lasciato un'importante testimonianza. Presidente, oltre a questo, devo dire che nella vita civile era un apprezzato avvocato penalista. Molti dei processi, che per tanti anni hanno occupato e segnato le cronache della nostra isola, lo hanno visto protagonista nel campo che gli apparteneva, come avvocato penalista di grande fama. grande fama. Esprimo il mio personale cordoglio alla moglie Lia, ai figli - Massimo e Roberto sono entrambi avvocati

Signor Presidente, ho appresso stamattina della morte del collega avvocato Mariano Delogu, cui ero legato da molti anni - da quando ho iniziato la professione - da una sincera e profonda amicizia oltre che una stima per le sue doti professionali e umane, che hanno contraddistinto tutta la sua carriera e la sua vita. Il collega Emilio Floris ha già descritto la figura del senatore Delogu: era una persona dalle doti umane straordinarie e oggettivamente fuori dal comune. Quando lo conobbi lui era già l'avvocato Delogu, una figura estremamente conosciuta protagonista di numerosissimi processi importanti nella storia dell'avvocatura sarda. Debbo dire che l'approccio con i colleghi più giovani era sempre caratterizzato da una grandissima umiltà e modestia, con una capacità di confronto che raramente si trovano nei colleghi, se non in quelli in possesso di doti profonde, come era appunto l'avvocato Delogu. ha ricoperto numerosi incarichi ed era una persona conosciuta e benvoluta da tutta la Sardegna, essendo stato anche presidente del Cagliari. È un uomo che ha dato davvero tanto alla Sardegna, allo sport e alla politica. È stato due volte sindaco di Cagliari: anche in quella circostanza ha saputo farsi apprezzare da tutti per la vicinanza

Ciò gli è stato riconosciuto, insieme alla grandissima correttezza nei confronti di tutti gli avversari, doti che facevano apprezzare, prima che il politico, l'uomo Mariano Delogu. Questo è stato ciò che ha contraddistinto sempre la sua vita. Credo di potermi unire alle manifestazioni di cordoglio, a nome anche di tutto il Gruppo del Partito Democratico, esprimendo la vicinanza ai familiari, alla moglie Lia e ai tre figli, in particolare a Massimo e a Roberto, ai quali sono personalmente legato da una profonda amicizia, perché anche con loro, entrambi avvocati, ho condiviso numerose battaglie nelle aule giudiziarie. La Sardegna perde una figura importante, che è stata un punto di riferimento per molta gente. Al di là della diversità delle opinioni politiche, quello che si si apprezzava nei confronti di quest'uomo era la sua umanità, la capacità di stare vicino alla gente e la capacità di confrontarsi. Vorrei ricordare anche un'altra dote dell'avvocato Delogu: una finissima ironia,

che denotano tanto l'umanità di cui ho già parlato, quanto quella finissima ironia che ha contraddistinto ogni sua azione. Riusciva a trovare l'aspetto simpatico anche nelle vicende più nelle vicende più serie e qualche volta drammatiche; riusciva sempre a portare con sé questa vena ironica. Pertanto, nel confermare la vicinanza a tutti i familiari, piango la scomparsa di un grande uomo e anche di un

il mio Gruppo parlamentare alle parole bellissime di Emilio Floris e di Giuseppe Cucca. Ci sarebbe da aggiungere poco, perché loro hanno conosciuto in prima persona

e, se mi consente, professionale. È stato un grande avvocato, un grande penalista, ed è stato un grande sportivo, con un enorme amore per la squadra della sua città, il Cagliari, di cui è stato anche presidente. È stato uno straordinario amministratore e credo che questo gli vada riconosciuto da tutte le parti politiche di quest'Aula, perché i sindaci di per sé, quando fanno bene il loro lavoro, penso che debbano avere un riconoscimento a 360 gradi. Non possiamo essere sempre viziati dalla politica; il giudizio politico è una cosa, ma il giudizio sulle amministrazioni è un'altra. Infine, è stato senatore. Probabilmente, di tutte le sue esperienze è quella che lo ha appagato di meno dal punto di vista personale, ma ha dato modo a tanti di noi di conoscerlo qui a Roma, nei banchi del Parlamento, del Senato e, per quanto mi riguarda, anche per fatti di carattere personale. Anch'io ho saputo questa mattina, nelle prime ore, della scomparsa di Mariano Delogu. Voglio dire che ha dimostrato nella sofferenza di questi mesi una grande voglia di vivere. È stato un combattente fino alla fine e non si è mai arreso, fino a quando la malattia non ha avuto il sopravvento. Credo che sia

*(PD)*. Signor Presidente, Mariano Delogu è stato una persona di parte, deciso ad affermare di esserlo sia nel suo ruolo di sindaco che di parlamentare. Lo voglio ricordare soprattutto nel suo ruolo di amministratore della mia città, Cagliari. Io ero il giovane segretario del maggior partito di opposizione della sua giunta, eppure ho sempre pensato e anche il mio partito ha sempre pensato a lui come ad un grande sindaco per Cagliari. Ho sempre apprezzato, in particolare, la sua ambizione di consegnare una città più moderna di quella che aveva trovato all'inizio del suo mandato (in questo recuperando le aspirazioni di grandi suoi predecessori, primo fra tutti Bacaredda) e la visione di una città a dimensione nazionale ed europea. A Delogu e alla sua giunta si deve l'inizio di un percorso che, nel corso degli anni (in verità pochi), ha permesso di riconsegnare ai cittadini spazi che per decenni erano stati tolti alla loro fruizione, la riqualificazione di interi quartieri storici e una rinnovata sensibilità cittadina alla cultura nelle sue varie forme. Noi lo chiamavamo, in maniera un po' spregiativa nel gioco delle parti politiche, "il sindaco dei giardinetti", ma a Delogu in realtà si deve una nuova, seria attenzione al recupero di spazi di ricreazione e di aggregazione - soprattutto di spazi verdi - per i cittadini di Cagliari. Una personalità forte che sapeva anche essere dura con i suoi avversari, ma certamente trasparente e libera, quindi degna di leale rispetto. La sua scomparsa è certamente una grande perdita per Cagliari e per la Sardegna tutta.

che con lui è iniziata a Cagliari, con le nuove modalità di elezione dei sindaci, una stagione

più di ogni altra cosa, quella funzione di primo cittadino, e che la funzione politica cui lui era più legato fosse quella del governo della sua città,

per quello che rappresentava in modo particolare il Cagliari nella Sardegna e per la città che esprimeva la squadra di calcio. Non si è mai allontanato neppure negli anni successivi da quella passione, che ha coltivato con grande impegno, con grande dedizione e anche con risultati importanti. Noi vogliamo ricordare Mariano Delogu per la sua efficienza e capacità di amministratore, per la sua qualità di impegno nella funzione politica e nella funzione professionale, ma anche come un cittadino